In data 30 dicembre 2021, è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della salute:* «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione

«Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»

nei giorni scorsi «Report» ha documentato la truffa dei diamanti (per 1,3 miliardi di euro), venduti a malcapitati correntisti al triplo del prezzo di mercato. Si tratta di una frode sulla quale hanno indagato l'Antitrust e nel 2017 la procura di Milano,

«Report» ha mandato in onda la testimonianza di un funzionario del *team* di ispettori di Banca d'Italia, Carlo Bertini, che ha rivelato il coinvolgimento dei massimi vertici di MPS nella truffa dei diamanti.

Bertini spiega che, mentre indagava su MPS, ha acquisito sufficiente documentazione da fargli sospettare un accordo tra Viola, Profumo e il *manager* di DPI, Maurizio Sacchi, nella vendita dei diamanti. Profumo e Viola, nel periodo di inizio della truffa dei diamanti, erano Presidente e amministratore delegato di MPS. Bertini, da retto funzionario, riferisce la *combine* al suo capo servizio di Banca d'Italia, Ciro Vacca: mossa incauta nel Paese alla rovescia, con onesti perseguitati e furbi senza scrupoli premiati. Qualcuno fa capire a Bertini che non è il caso di alzare un polverone: vuoi stare tranquillo o vuoi partire con una guerra? Contro chi? Bertini porta le sue rimostranze sul tavolo del capo della vigilanza Paolo Angelino, il quale ribatte:

«Report» ha documentato il coinvolgimento nel *business* dei diamanti di politici, avvocati e massoni legati alla 'ndrangheta. Quando Bertini scopre i presunti legami che ruotano intorno a Pittelli, segnala al vice direttore generale di Banca d'Italia Perrazzelli, che gli risponde: "gestire questo tipo di cose richiede una grande libertà; non mi sembra che sia la modalità non solo qua dentro, ma in tutte le grandi strutture, che si muovono in maniera militare; nella mia vita professionale, mi sono trovata di fronte a cose spaventose, nei confronti delle quali mi veniva detto che dovevo essere come una statua di marmo, quindi farmele scivolare addosso come l'acqua e questa cosa qui mi ha aperto gli occhi su come in Italia e nel mondo si fa carriera". Invita dunque Bertini a farsi scivolare addosso la vicenda e chiudere non un solo occhio, ma tutti e due. Signor Presidente, in conclusione, è uno scandalo che vede coinvolti i massimi vertici di Banca d'Italia e mai documentato prima, il quale apre un varco nella cortina di omertà, protezione istituzionale e servile obbedienza alla gerarchia e spiega la complicità della vigilanza nei *crack* e dissesti bancari, con almeno un milione di famiglie frodate dalle bancarotte seriali degli ultimi anni, per un valore stimato di 200 miliardi di euro. Ho presentato sul tema un'interrogazione, cui mi auguro che il Governo risponderà.

In altre parole, il Parlamento non ha ancora potuto esprimersi sul decreto-legge del 26 novembre, che piovono quelli del 24 e del 30 dicembre e ora i *mass media* di regime stanno preparando la strada per un ulteriore, pauroso decreto, con misure allucinanti, che viene annunciato per il 5 o il 7 gennaio. Questo nella totale impossibilità del Parlamento di dire la sua, persino su quello del 26 novembre, ampiamente superato da tutte le misure che vengono giorno per giorno introdotte, auspicate e imposte attraverso attraverso i *media*, quando Paesi che hanno maggiore rispetto per la loro Costituzione, che pure non è scritta (come nel caso del Regno Unito), stanno abolendo le poche restrizioni che avevano. A questo si aggiungono i Ministri che mentono: il ministro Speranza mente qui in Aula sul suo interessamento per bloccare l'indagine dell'Organizzazione mondiale della sanità; il ministro Lamorgese mente in Commissione, dicendo che non è vero che i poliziotti vengono sospesi dallo stipendio, anche se assenti o in gravidanza.

mancata risposta a tutte le interrogazioni su tutte le questioni Covid. Ne ho presentata una proprio adesso sul fatto che, da indagini sia del Regno Unito sia della Danimarca (quella della Danimarca particolarmente importante, perché fatta sui dati dell'intera popolazione, e quella del Regno Unito basata sui dati ufficiali dell'agenzia per la salute di quel Paese), emerge che i vaccini, dopo un certo periodo, hanno una efficacia negativa. negativa. Qui c'è un medico, che ringrazio per essere presente come rappresentante del Governo (è insolita la presenza di un rappresentante del Governo in una seduta come questa): "efficacia negativa" dovrebbe far tremare le mani a chi si accinge a votare ulteriori obblighi di questo tipo. Chiedo al Governo di ricordarsi che c'è una Costituzione, che c'è un Parlamento e che c'è la salute dei cittadini di mezzo. Non si può scherzare, non si possono fare forzature.

La seduta è tolta